"Il link apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 21 dicembre 2012 Onorevole Presidente, La informo che in data odierna, tenuto conto della situazione politica venutasi a determinare, ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni del Gabinetto da me presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto e ha invitato

SENTITI i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; decreta Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma il 22 dicembre 2012 *F.to* Giorgio Napolitano». **Sui lavori per effetto dello scioglimento delle Camere, 1'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari. Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo. Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta. Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa qualunque ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati. Infine, il regime di *prorogatio* del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento di atti relativi agli *interna corporis* dell'Assemblea.

Segnalo che, nonostante si siano diffuse notizie diverse, l'aggiornamento delle tabelle relative ai deputati e ai senatori eleggibili sulla base del censimento del cambia esclusivamente la classe delle firme per il Trentino-Alto Adige, che avendo superato un milione di residenti slitta dalla seconda alla terza fascia. Com'è noto, questo tipo di decretazione è ammissibile, perché non si tratta della materia elettorale, identificata dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, poi richiamata dalla legge n. che si riferisce esclusivamente al «nucleo duro» del sistema, alla formula elettorale, cioè alla trasformazione dei voti in seggi. Qui siamo esclusivamente nell'ambito della legislazione di contorno, che pure è molto importante in termini di *standard* democratici. L'esigenza del decreto-legge è emersa a causa del nostro fallimento in materia di riforma elettorale. Un fallimento collettivo, di cui dovremo fare memoria, anche per evitare che si riproduca nella legislatura prossima. Va probabilmente fatto un ragionamento più serio su quando approvare le riforme elettorali e anche le riforme della legislazione di contorno. Non è vero che bisogna farle a fine legislatura, come teorizza una parte della dottrina, perché altrimenti il Parlamento sarebbe delegittimato. È delegittimato nella sua forza quel Parlamento che invece non riesce tempestivamente a fare queste riforme. Pertanto, il tema della riforma elettorale dovrebbe essere ripreso all'inizio della prossima legislatura, potendo contare su un velo di ignoranza dei rapporti di forza nelle elezioni successive. Altrimenti rientriamo nel gioco di previsioni, sondaggi e altro, che rende difficile un'intesa effettiva, perché tutti vivono questo momento come un gioco a somma zero. In quella sede bisognerà anche valutare attentamente tutti gli aspetti deficitari - e sono molti - del procedimento elettorale. C'è un lavoro di ammodernamento del procedimento elettorale, al di là della formula,

si è stati costretti a intervenire in questa materia con decretazione, il che rende problematico il percorso perché le norme elettorali dovrebbero essere fisse dovrebbero essere fisse e largamente prevedibili per tempo. Il Governo si era incaricato, soprattutto rispetto alla raccolta firme, di emanare questo decreto, che presentava qualche incongruenza interna, che per nostra fortuna è stata sanata dalla Camera dei deputati, riconducendolo a razionalità. pertanto, altamente opportuno che oggi noi lo approviamo in via definitiva e garantiamo che, a partire dalla raccolta delle firme, la competizione verso le elezioni avvenga in modo ordinato. Restano i problemi sottolineati anche dai colleghi radicali, ma quelli dovranno essere risolti a regime. Sarà importante che la prossima legislatura li affronti sin dall'inizio*. intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia‑Centrodestra Nazionale al provvedimento, alla luce del fatto che, approvandolo, si metteranno tutti i movimenti e i partiti in grado di partecipare in maniera equa alla competizione e alla consultazione elettorale.

Si stava per procedere ad approvare una norma che, a stretto rigore, necessitava della maggioranza assoluta dei presenti in Aula assolutamente disinteressandosi del fatto che la settimana scorsa fosse o meno presente in Aula la maggioranza necessaria Normalmente, proprio perché trattasi di decretazione su materia elettorale, il Governo coinvolge tutte le forze politiche, maggioranza e opposizioni. Così non è stato. Il Governo non ha fatto un buon servizio, ha fatto di testa sua e ha calato sull'Assemblea

di approdare in Parlamento. Così non è, così non sarà e così non vogliamo che si possa leggere. Pertanto, a nome della Lega, annuncio la nostra astensione.

alla Camera dei deputati per consentire che sia i soggetti esterni non presenti in Parlamento, sia quelli già presenti in Parlamento possano partecipare alle elezioni in condizioni di equilibrio e, anzi, di parità. Mi sembra che nei tempi ristretti che sono richiesti per la raccolta delle firme e per la partecipazione alle elezioni la soluzione definita dal Parlamento sia corretta ed equilibrata. *(Applausi

e dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell' interno*: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» Il provvedimento è stato assegnato alla la Commissione permanente per l'esame dei presupposti di costituzionalità, nonché alle Commissioni permanenti riunite 3a e 4a, in sede referente, con i pareri delle Commissioni la, 2a, 5a, 6a e 14a.

nella votazione sul disegno di legge n. 3647, pur essendo presente in Aula, per mia imperdonabile distrazione non ho votato. Vorrei che risultasse agli atti la mia presenza e che ovviamente avrei votato favorevolmente.